Spadoni Urbani, Germontani, Blazina, Marinaro ed i senatori, un po' meno numerosi a dire il vero, Di Giovan Paolo, Malan, Pedica e Possa. Mi scuso anticipatamente se la mia replica non sarà esaustiva né completamente organica, ma le questioni poste sono molte, anche molto differenti tra loro, e tutte egualmente importanti e meritevoli almeno di un tentativo di risposta. I primi interventi sono stati tutti focalizzati sulle politiche di parità e sul recepimento della direttiva n. 54 del 2006. I dati già elencati dalla senatrice Bianconi in materia di occupazione femminile sono effettivamente sconfortanti. Questa è veramente l'ennesima direttiva sulla parità e le pari opportunità che ci apprestiamo a recepire e credo di poter condividere appieno molte delle cose dette dalle senatrici intervenute. Già moltissime volte in quest'Aula abbiamo discusso di parità, di politiche di conciliazione, di reale possibilità per le donne, che sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese, di fare pienamente la loro parte.

paradossalmente rischia, all'interno della nostra società, di diventare il limite della nostra azione. La nostra società deve cambiare culturalmente e capire che i problemi delle donne non sono solo delle donne, ma sono delle donne e degli uomini, che insieme devono trovare le soluzioni.

sono conscia che esiste una sentenza della Corte europea, ma sono convinta che si tratti di un tema sul quale debba esserci ampio confronto da parte del Governo, di tutti i Ministri interessati, con le parti sociali e con l'Europa,

Certo è che per le donne non deve derivare alcuna penalizzazione dall'adempimento della sentenza: giusto parlare del problema, ma questo non deve destabilizzare e rendere ancora meno sicure le donne, e in generale le persone, del loro futuro, specialmente in un momento di crisi e di insicurezza come questo. Ritengo pertanto auspicabile e preferibile non cercare ora soluzioni affrettate all'interno di questo provvedimento.

per aver rimarcato, come pure la senatrice Marinaro, la necessità di modificare il Regolamento del Senato in modo tale da poter esaminare la legge comunitaria in un momento distinto dalla Relazione. La senatrice Marinaro ha fatto poi un accenno all'utilizzo dei fondi europei, argomento cruciale sul quale la 14a Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva, che credo sarà completata per l'estate e che potrà essere una base di discussione importante. La senatrice Marinaro ha anche sollevato il problema della necessità di copertura quando il recepimento delle direttive comunitarie avviene per delega; è un argomento interessante che penso sia degno di essere seriamente discusso all'interno della Commissione bilancio. Senatore Malan, è vero, il diritto comunitario sta diventando veramente pletorico e si dovrebbe tendere alla semplificazione per non appesantire i cittadini europei e renderli sempre più insofferenti verso un'entità che spesso percepiscono solo come un peso burocratico. Mi viene spesso da domandare se veramente il principio di sussidiarietà sia applicato nelle direttive e penso che dobbiamo, come ho già detto nella relazione iniziale, lavorare molto di più nella fase ascendente dei provvedimenti. Senatore Pedica, che siano entrate disposizioni estranee non lo credo possibile, data la severità delle norme regolamentari con cui viene gestita la comunitaria;

delle sentenze di condanna definitive, la ritengo veramente uno strumento indispensabile, certo dovrà essere recepita dagli altri Paesi. Voglio fare però una precisazione: in particolare con la Romania, esiste un accordo quadro bilaterale, già dal 2003. Lei sa che proprio ad una delegazione di parlamentari romeni che è venuta in Commissione abbiamo fatto notare che non si stanno dando molto da fare per applicare quella decisione quadro; spero dunque che siano più veloci nel recepire la direttiva, in maniera tale da poter lavorare al meglio.

ascoltato in audizione - come regolarmente fa presso la Commissione - ha chiarito che la questione di Rete4 non è oggetto di procedura d'infrazione. La sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 31 gennaio 2008 si inquadra, invece, in un procedimento pregiudiziale, in cui il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte una sentenza di interpretazione di una norma comunitaria in materia di risarcimento. dovesse ritenere che tale sentenza non sia stata adempiuta, potrebbe allora decidere di aprire una procedura d'infrazione, che però, per il momento, non esiste. Riguardo alla direttiva sui rimpatri, forse avrà notato che ho presentato a mio nome un emendamento soppressivo, proprio perché si tratta di una direttiva molto complicata: così com'è, non sono stati specificati principi e criteri di delega, richiede il concerto di numerose amministrazioni dello Stato, quindi è preferibile non rimandarla chissà di quanto, bensì corredarla appunto dei criteri e principi di delega. Senatore Possa, sono anch'io molto preoccupata per la direttiva servizi, perché credo che sarà una rivoluzione, per come siamo abituati noi e per com'è abituata a lavorare la pubblica amministrazione. Condivido tutte le sue osservazioni riguardo la sicurezza, la qualità dei manufatti e così via: purtroppo, però, tra gli aspetti che prevede la direttiva c'è proprio quello di non poter richiedere come requisito la reciprocità; quindi, questo purtroppo non si può fare. Credo che bisognerà seguire molto da vicino l'emanazione del decreto legislativo corrispondente, in maniera tale da lavorare al meglio.

finestra"). Il Senato della Repubblica, esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.*

Signora Presidente, onorevoli relatrici, onorevoli senatori, la legge comunitaria 2008 giunge all'esame dell'Aula Commissione - abbastanza travagliato, in primo luogo, a causa all'interruzione anticipata della legislatura e alla conseguente necessità, da parte del nostro Governo, di ripresentare e riproporre Questo inevitabile ritardo ha finito per mettere in luce lo sfasamento esistente tra i dati contenuti nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferiti al 2007 e quelli riferiti all'epoca in cui essi vengono all'esame di questo Parlamento.

Su questo punto devo dire che condivido le preoccupazioni della relatrice, senatrice Licastro Scardino: abbiamo infatti allo studio la possibilità di separare nei tempi la discussione della Relazione dalla presentazione del disegno di legge comunitaria annuale. Questa separazione temporale potrà costituire, secondo noi, l'occasione per confrontarsi più volte all'anno sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e sulla opportunità profonda che si possano aprire in questo contesto importanti spazi per gli interessi nazionali. Credo sia necessario, voglio ricordarlo con l'amico senatore Di Giovan Paolo, proprio in quest'anno in cui andiamo verso le elezioni europee (si voterà tra qualche settimana), uno sforzo comune di tutte le istituzioni affinché l'Europa sia percepita dai cittadini non solo come un fastidioso vincolo, ma soprattutto come un'occasione di sviluppo e di crescita democratica. Colleghi senatori, vorrei, a margine di questo mio intervento, fare una considerazione: credo che lo sforzo di tutti sia quello di lavorare per disegnare una nuova concezione di Europa;

che costringe a parlare soltanto di bollini e argomenti simili, mentre in questo momento l'Europa ha bisogno di anima, ha bisogno di una partecipazione forte, ha bisogno di occuparsi dei grandi problemi, come la grande crisi economica, la sicurezza, il lavoro,

In questo quadro, ritengo che un'azione particolare debba essere riservata alla fase cosiddetta discendente, proprio in vista della tutela degli interessi nazionali nella fase ascendente. Sono persuaso che la rafforzata partecipazione a questa fase da parte del Parlamento italiano e dei Parlamenti nazionali contribuirà notevolmente a fare emergere la nostra idea di Europa, alla quale facevo prima riferimento. Venendo al merito del disegno di legge, desidero innanzitutto ringraziare

il primo approccio ad un grande ragionamento che tutti insieme dobbiamo fare sull'Europa. Nel corso della discussione generale, molti sono stati gli interventi di senatrici che hanno posto l'attenzione sul tema della parità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, oggetto di una delle direttive contenute nella legge comunitaria, e hanno richiamato il Governo all'impegno per dare attuazione alla ormai tanto declamata e famosa recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

sempre con uno sguardo attento ad una grande crisi economica che, in queste ore e in questi mesi, sta colpendo le fasce più povere e più deboli della nostra società. Non è ancora maturata una decisione sullo strumento legislativo che dovremo utilizzare, né sui tempi dell'intervento; per questa ragione non posso impegnare, alla luce anche di quello che ho appena detto, il Governo rispetto a scelte che dovranno essere assunte collegialmente. Voglio ribadire che l'impegno del Governo su questo l'impegno del Governo su questo tema, ne abbiamo parlato più volte, è quello di aprire una larga consultazione con le parti sociali, con i sindacati, con tutte quelle forze economiche e produttive del Paese che, senza pregiudizio ideologico, vorranno su questo tema aiutare il Governo e le parti sociali non soltanto a rispondere ad una richiesta dell'Europa, ma, come ho detto prima, ad invertire una rotta e far sì che questa sia un'occasione per riscrivere una vera, seria, grande politica per la famiglia.

poi grato alla presidente Boldi per aver ricordato l'emendamento del Governo volto ad anticipare il recepimento di quella famosa ed importante decisione quadro, adottata il 27 novembre dello scorso anno, in base alla quale le sentenze di condanna pronunciate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato, potranno essere scontate nel Paese d'origine. Se vogliamo restituire la percezione della sicurezza ai nostri cittadini ed evitare che nascano orribili spinte xenofobe o razziste nel nostro continente e nella nostra Nazione,

senatore Pedica voglio ricordare, come ho già detto in Commissione, che la decisione di anticipare il recepimento è stata accompagnata da iniziative diplomatiche in tal senso. Ricordo all'Assemblea

prigioni. Quanto alla restante parte dell'articolato, mi limito per brevità a citare la direttiva servizi che, come è stato ricordato, sarà una fondamentale occasione di apertura del mercato interno e di semplificazione amministrativa. Sono d'accordo poi con quanto detto dal senatore Di Giovan Paolo, che ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento della 14a Commissione nei lavori del Senato, perché l'esperienza di questi giorni ci dimostra che problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario si pongono

sul cosiddetto regolamento della TV dei minori. Preannuncio che noi respingeremo qualsiasi tipo di ragionamento, ma voglio impegnarmi, a nome del Governo e non solo personalmente, perché perché chi vi parla, così come l'intero Governo, sarà attentissimo e non consentirà alcun tipo di transizione su un tema che ci vede impegnati moralmente, prima che politicamente, quello cioè della difesa dei minori e della tutela dell'infanzia, rispetto ad un mercato televisivo

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 144-*bis,* commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, ovvero che non siano stati respinti in sede di Commissione o non si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa. Pertanto, ai sensi delle richiamate norme regolamentari, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti:

nonché 20.0.400 e 24.0.200 del Governo.

1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che: all'articolo 9, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, al comma 5, si si escluda che gli adempimenti previsti siano a carico anche delle amministrazioni regionali, considerando peraltro che la disposizione in esame reca una delega legislativa; - all'articolo 15, all'articolo 15, la clausola di salvaguardia, di cui al comma 13, non contenga norme di carattere imperativo dirette alle Regioni e alle Province autonome; - all'articolo 18, si escluda l'obbligo, anche in capo alle Regioni e alle Province autonome, di adoperarsi per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici a livelli corrispondenti alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, potendo ciò rappresentare una limitazione dell'autonomia regionale e locale. Quanto all'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria, si osserva che la disposizione abrogatrice, di cui al comma 1, lettera potrà essere attuata nel presupposto che le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive siano disposizioni di legge statale, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire. Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sugli identici emendamenti 9.200 e 9.201, nonché sugli identici emendamenti 9.202 e 9.203, parere non ostativo, osservando che le disposizioni ivi previste possono comportare una violazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e agli enti locali in materia di micro e piccole imprese, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'attività imprenditoriale; sull'emendamento 11.202, parere non ostativo, osservando che il criterio di delega di cui al capoverso 1-*bis*, lettera dal momento che prevede azioni specifiche finalizzate alla diffusione dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, potrebbe determinare una indebita limitazione delle competenze regionali e locali in materia;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.200, 41.207, 11.104, 11.103, 11.106, 24.202 e 11.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 11.202, 15.200 15.201, sulle quali il parere è di contrarietà semplice. Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 43.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 5 sia sostituito dal seguente: Alle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Presidente, relativamente ai pareri testé letti, volevo sottolineare all'attenzione del Governo e della relatrice che c'è un parere della Commissione affari costituzionali abbastanza puntuale e condizionato. Infatti, la 1a Commissione non esprime parere favorevole, se non saranno modificate alcune parti del testo; naturalmente, si tratta di lievissime modifiche, che sono però lesive delle competenze regionali. Si tratta di due o tre punti. Siccome c'è una

queste parti che contrastano con l'articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda i poteri statali e regionali, così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.

con l'emendamento 3.2 ci proponiamo di ricordare la necessità di ottemperare, nell'esecuzione della delega, anche al principio di sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive. L'emendamento

che trovano la loro origine spesso nel fatto che per un periodo indefinito restano vive, soprattutto nel caso di direttive autoapplicative...

le vostre conversazioni fuori dall'Aula. Diventa anche antipatico per il vice Presidente di turno continuare a scampanellare. Prego, senatrice Dicevo che ci troviamo di fronte ad un numero molto alto di infrazioni e di contenziosi che derivano dal fatto che, soprattutto nel caso delle direttive autoesecutive,

Quindi, anche la predisposizione delle necessarie regolamentazioni delle misure di infrazione e di pene amministrative pecuniarie e quant'altro deve prevedere da parte delle istituzioni della Repubblica, siano esse quelle nazionali o quelle locali, una procedura di adeguamento chiara, trasparente e tempestiva.

aggiuntivo. Pregherei i colleghi di prestare attenzione perché quest'emendamento non entra nel merito di singole politiche o di aspetti particolari, pure importanti, ma riguarda la procedura Come i colleghi sanno, noi votiamo, affrontiamo e discutiamo contemporaneamente la relazione del Governo e la legge comunitaria.

il Parlamento non discute quell'atto che sarebbe il più qualificante per lo svolgimento del proprio ruolo, cioè la relazione. stesso tempo il consuntivo dell'anno precedente ma anche l'individuazione di punti critici e di proposte che vengono, o dovrebbero, essere indirizzate

per interloquire direttamente con gli organi comunitari? Quale altro momento ha il Parlamento per esercitare la sua funzione principale in questa materia, che è quella di indirizzo o, per usare un'espressione comunitaria ed europea, per intervenire nella fase ascendente, contribuendo quindi al formarsi delle normative comunitarie? È inutile poi che tutti ci lamentiamo quando giunge la direttiva, che viene vissuta in qualche modo come estranea, come un elemento che si sovrappone in modo estraneo alla normativa nazionale, se noi stessi non esercitiamo la nostra funzione,

di separare i due momenti per esaltare e dare concreta possibilità al Parlamento di esercitare il suo ruolo.

per incoraggiare la revisione del Regolamento del Senato - come abbiamo detto tutti stamattina - è sicuramente condivisibile, ma se fosse approvato così com'è, si otterrebbe l'effetto perverso che, nel caso la modifica del Regolamento del Senato non passasse celermente,

Signora Presidente, mi permetta di chiosare brevemente l'opinione espressa sia dalla relatrice che dal Ministro. Quando si apprezza così tanto il contributo di un senatore di opposizione si cerca di accoglierlo.

Magari si trovi una formulazione, mi si inviti a trasformarlo in un ordine del giorno, si dia un segno d'interesse per il fatto che ho sollevato, anzi, che abbiamo sollevato una questione importante e condivisa. Chiudo la parentesi.

del nostro Governo, che magari giustamente si è opposto in qualche modo ed ha subito un'infrazione, ma il conforto del Parlamento non può essere *a**posteriori*, ci deve essere un coinvolgimento immediato nella formazione dell'opinione del Parlamento stesso e quindi dell'indirizzo su come e se ci si deve opporre ad un'infrazione. Ad esempio, per l'infrazione sul pensionamento non abbiamo visto un'opposizione così forte come l'abbiamo vista invece in settori che riguardavano il sistema radiotelevisivo italiano.

(testo 2) è motivato dalla necessità di riordinare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 193 del 2007, di attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE, relativa al regime sanzionatorio sui controlli in materia di sicurezza alimentare. Nel disposto non si tiene conto che il regolamento (CE) 852/2004 prevede una certa flessibilità nelle procedure di autocontrollo per le micro e piccole imprese, riconfermata nelle linee guida comunitarie sulla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP. In queste imprese, infatti, il regolamento sopra accennato stabilisce che non sempre è possibile identificare i punti critici di controllo e la buona prassi può sostituire la sorveglianza dei punti critici. I documenti e le registrazioni sono adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa ed è possibile derogare all'allegato secondo il regolamento. L'atteggiamento del legislatore, invece, è stato quello di reintrodurre il principio della sanzione preventiva, con aggravamento dei livelli sanzionatori a discapito della prescrizione *a* *priori* che era stata prevista quale criterio fondamentale nei principi dell'autocontrollo

una maggiore consapevolezza degli operatori alla collaborazione con le autorità di controllo, contribuendo al miglioramento dei livelli di sicurezza delle produzioni alimentari, con forti riduzioni, se non la quasi scomparsa, di casi di tossinfezioni.

(testo 2) e tende sostanzialmente a facilitare la vita al mondo delle piccole e medie imprese che operano nel settore alimentare, tenendo conto del fatto che la normativa comunitaria, così come introdotta dalla direttiva europea 2004/41/CE è stata recepita dal decreto legislativo n. 193 del 2007 in maniera disarticolata rispetto al contenuto del cosiddetto pacchetto igiene che è composto da una serie di regolamenti comunitari immediatamente applicabili nel nostro ordinamento e di cui si parla all'articolo 9. Questi regolamenti hanno introdotto un principio fondamentale che è quello dell'autocontrollo dell'operatore del settore alimentare, che si responsabilizza nel porre in essere una serie di pratiche consistenti nel raggiungere l'obiettivo della sicurezza alimentare.

nella produzione alimentare, in quanto, anziché rafforzare il concetto di autoresponsabilizzazione dell'operatore alimentare, si ritiene di dover provvedere con controlli preventivi e con un meccanismo sanzionatorio che ne impedisce una corretta modalità di svolgimento in conformità alla normativa comunitaria.

con molta retorica e passione, cioè l'impegno del Governo per quanto riguarda le pari opportunità e le donne. Siamo in presenza di una direttiva ad una fusione delle sette direttive precedenti, adottate in anni diversi, che però, a livello italiano, riscontrano delle difficoltà di piena applicazione. Con questo emendamento vogliamo soltanto verificare e soprattutto impegnare il Governo a procedere alla emanazione del decreto, non all'adozione, entro il 15 agosto 2009. Così credo che possiamo verificare, tenendo conto della situazione particolare del nostro Paese, una crisi così profonda che tocca in particolar modo le donne, quale è il grado di impegno del Governo a fare in modo che il decreto applicativo di questa direttiva sia emanato entro il 15 agosto 2009.

11.200. All'articolo 11 la data del 15 agosto 2009 è posta con riferimento all'adozione del decreto legislativo, stabilisce il termine ultimo del 15 agosto per l'entrata in vigore dell'atto di recepimento. Con questo emendamento proposto si vuole sanare una potenziale inadempienza da parte dello Stato italiano in quanto, data la tempistica che intercorre tra l'adozione del decreto e l'emanazione dello stesso, il decreto potrebbe non entrare in vigore nei tempi stabiliti dalla direttiva. Si ritiene invece doveroso adempiere al recepimento nei tempi fissati dal provvedimento comunitario, considerando che l'Italia si è già avvalsa della proroga di un anno concessa all'articolo 33 della direttiva. Ricordo a tutti che la proroga è concessa a quei Paesi che, come afferma la direttiva, presentino particolari difficoltà nel garantire la parità fra uomini e donne, e certo non è un messaggio positivo avvalersi della proroga per tutte quelle donne italiane che, ad oggi, subiscono discriminazioni sociali ed economiche nel mercato del lavoro, un livello di occupazione bassissimo rispetto alla media dell'Unione europea e il gravame delle cure familiari a loro carico. L'anno di proroga, colleghi signor Ministro, potrebbe essere impiegato in maniera fattiva e propositiva, adoperandosi per produrre ricerche di settore specifiche sulla condizione femminile, le quali al momento mancano totalmente, al fine di individuare quali azioni concrete, oltre l'enunciazione del principio delle pari opportunità, possano essere intraprese per rendere davvero sostanziale il diritto alla parità del trattamento.

ma già con questo emendamento si impone al Governo di rispettare almeno il termine di un anno della proroga senza rischiare di oltrepassare anche questo.

che il Governo deve mettere in campo per realizzare effettive condizioni di parità nel nostro Paese fra gli uomini e le donne. fin da subito, l'indicazione dell'adozione di un fondo speciale di investimento finalizzato a queste azioni positive. Riteniamo che la parità costi e che sulla parità si debba investire. Il fondo deve essere finalizzato a garantire innanzi tutto misure incentivanti per il lavoro, anche di natura fiscale. Stamattina la collega Bianconi ha ben richiamato i dati sul *gap* occupazionale che riguarda il nostro Paese*,* un *gap* di genere. Voglio ricordare il fatto che questi dati così sconfortanti rischiano di essere pesantemente peggiorati dalla crisi in atto. I dati resi una settimana fa dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) dicono che le donne pagheranno la crisi con un peggioramento della propria condizione occupazionale di almeno dieci punti superiore a quello degli uomini. Inoltre, riteniamo che debbano essere destinate risorse specifiche a superare gli svantaggi di carriera, intesi come accesso ai posti di lavoro maggiormente qualificati e come accesso accesso alla rappresentanza. Ricordo che in Italia le donne ai vertici aziendali sono solo il 4 per cento dei rappresentanti dei *board* aziendali e che anche in questo Parlamento il differenziale di rappresentanza è pesantissimo: abbiamo solo il 18 per cento di parlamentari donne, a fronte del 21,7 per cento, pur basso, dell'Unione europea. Ancora, crediamo si debbano destinare risorse specifiche per garantire l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, sia in termini di reddito che di previdenza (parliamo in questo caso di contribuzione figurativa), figurativa), di congedi, di flessibilità organizzativa del lavoro e di reimpiego delle donne che rientrano da periodi di cura, come elemento di diritto, di prevenzione di ogni discriminazione, come condizione essenziale per l'esercizio effettivo della parità lavorativa, ma anche come sostegno alla natalità del nostro Paese. Ricordo che il 15 per cento delle donne già occupate subisce pesanti peggioramenti della propria condizione lavorativa o perde il lavoro a seguito dell'assenza per maternità. Chiediamo poi di finalizzare risorse all'attuazione di un piano straordinario di servizi di cura, rivolti all'infanzia e alla non autosufficienza, condizioni che sono al centro degli impegni di cura di tutte le donne nel corso della propria vita. Vale ricordare un dato purtroppo noto: i servizi all'infanzia in Italia si fermano ad un'offerta del 12.3 per cento, a fronte fissato dalla strategia di Lisbona; e manca ancora la determinazione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni per le persone non autosufficienti, previsti dalla legge n. 328 del 2000; non è infine stato adeguato il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Tutti questi investimenti sono indispensabili per garantire che le energie delle donne possano essere destinate al lavoro retribuito e non prioritariamente a quello di cura. Infine, voglio richiamare il fatto che - in coerenza con il dettato dell'articolo 141 del Trattato di Lisbona, richiamato dall'articolo 14 della direttiva di cui

che purtroppo - com'è noto - danno luogo all'inqualificabile fenomeno delle dimissioni in bianco. Da ultimo, con lo scopo che effettivamente non avvengano discriminazioni ed organismi pubblici possano vigilare in maniera efficace sull'eliminazione delle discriminazioni di genere, chiediamo che alle commissioni regionali di parità vengano affidate tutte le funzioni previste dall'articolo 20 della direttiva. queste richieste finalizziamo una dotazione di risorse importante, ma che riteniamo minima e indispensabile per ottenere gli obiettivi di parità richiamati: parliamo di parliamo di 1,2 miliardi di euro all'anno per tre anni, che potranno migliorare le condizioni di lavoro di milioni di donne e produrre nuova occupazione, migliorando anche gli indici economici del nostro Paese. Ricordo che per 100.000 nuovi posti di lavoro destinati alle donne, si aumenta un quarto di punto del PIL: questo dà, di per sé, precisa idea del fatto che l'investimento operato in materia di parità occupazionale e di pari opportunità di genere rientra in termini di miglioramento della *performance* economica del Paese. La realizzazione delle condizioni alle quali finalizziamo questo investimento costituisce quindi presupposto di base preliminare per il raggiungimento della parità effettiva. Il loro soddisfacimento è, a nostro modo di vedere, condizione preliminare per l'esercizio della parità in ogni momento della vita lavorativa delle donne. Solo la preventiva e contestuale soddisfazione di queste condizioni Solo la preventiva e contestuale soddisfazione di queste condizioni potrà consentire di avviare un discorso più complessivo sulle condizioni di parità lavorativa fra i generi, ivi comprese le questioni che riguardano il trattamento previdenziale e l'età di accesso alla pensione,